riguardano lo stesso argomento. Nel merito, mi preme intanto sottolineare che parliamo di un'arteria strategica che collega Lecco alla Valtellina, la strada statale 36 «Del Lago di Como e dello Spluga», nel tratto tra Lecco e Colico, costruita tra gli anni '60 e la fine degli anni '80. Il tracciato che si sviluppa per circa 50 chilometri è importante, attraversa una serie ininterrotta di gallerie, anche di notevole lunghezza, e necessita quindi da sempre di imponenti attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Devo precisare che, come per tutte le opere di sua competenza, ANAS ci riferisce che provvede ad effettuare controlli periodici, per constatare l'effettiva sicurezza per l'utenza stradale. I numerosi interventi manutentivi effettuati da ANAS nel corso degli anni sulla statale 36 hanno interessato, tra l'altro, anche le canne di monte e valle della galleria Monte Piazzo, che, attraversando l'omonima montagna, situata all'interno di una faglia di carattere regionale, sono state oggetto di importanti effetti deformanti sin dall'originaria apertura al traffico della galleria stessa. E qui ci riserviamo di accertare anche le fasi di cantierizzazione dell'opera.

la circolazione dell'acqua che grava sulle strutture portanti, ANAS ha progettato lavori di consolidamento del contorno roccioso e di rifacimento del rivestimento dissestato della canna di monte (dal chilometro 84,485 al chilometro 84,905) e della canna di valle (dal chilometro 84,243 al chilometro 84,474), 84,474), della galleria Monte Piazzo, per un'estensione di circa 425 metri, lungo la canna nord, e per 231 metri lungo la canna sud. Nell'ambito di tale progetto, ANAS ha predisposto un dettagliato studio delle fasi relative alla chiusura alternata delle due canne e sono stati valutati gli effetti e i possibili disagi del cantiere sulla circolazione della strada statale 36. A tal fine, prima dell'avvio dei lavori, si sono svolte diverse riunioni con le prefetture e le amministrazioni provinciali di Lecco e Sondrio, dove sono state concordate e condivise le modalità di attuazione delle fasi operative. In particolare, per tutta la durata dei lavori, si è stabilito di mantenere la circolazione lungo la strada statale 36 in direzione Lecco, verso sud, su due corsie, a partire dalle ore 15-16 e fino alle ore 24 di ogni domenica, e di deviare, invece, il traffico in direzione Colico, verso nord, sulla strada provinciale 72. I lavori sono stati consegnati e avviati nel mese di giugno 2012, con la realizzazione del *by-pass* di Corenno e la centinatura di un tratto della canna di monte dal chilometro 84,285 al chilometro 84,485. Tale intervento, non previsto nell'originario contratto d'appalto dei lavori, è divenuto indispensabile a causa del manifestarsi di importanti lesioni alle strutture portanti della galleria. I lavori sono poi proseguiti dal mese di settembre 2012 con interventi nella canna di valle, attraverso il rifacimento delle strutture portanti della galleria, per circa 231 metri (in particolare il rivestimento in cemento armato dello spessore di un metro su tutto il contorno), su tutto il contorno), necessario per sostituire i tratti deteriorati risalenti all'epoca della costruzione del *tunnel*. Relativamente alla situazione deformativa sopra descritta e alle potenziali vibrazioni indotte dalle adiacenti lavorazioni di scavo, la canna di monte, in esercizio a doppio senso di marcia, è stata oggetto di un approfondito monitoraggio dal mese di settembre 2012. In particolare, le strutture sono state sottoposte a ispezioni visive, misure con fessurimetri, con martinetti piatti e con stazioni di convergenza. L'attività di monitoraggio da parte di ANAS ha consentito infatti di valutare compiutamente le variazioni degli stati tensionali e deformativi collegati alle intense precipitazioni piovose che, com'è noto, si sono abbattute sulla Lombardia dallo scorso mese di febbraio e che, di conseguenza, hanno incrementato gli effetti delle spinte idrauliche sulle strutture della galleria Monte Piazzo. Le letture effettuate in data 27 aprile 2013, pur indicando una progressione delle tensioni nel calcestruzzo del rivestimento, non avevano evidenziato l'insorgere di situazioni di criticità. Il 9 maggio scorso, invece, i controlli tecnici hanno fatto emergere alcune anomalie strutturali, amplificate, il giorno successivo, dall'incremento delle spinte gravanti sul rivestimento della galleria. Pertanto, il 10 maggio (quindi il giorno successivo) ANAS ha dovuto provvedere alla chiusura del traffico lungo la canna in direzione Nord della galleria. Ciò premesso, l'evento sopra descritto va senz'altro inquadrato nell'ambito dell'imprevedibilità. L'esame delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati e descritti poco fa ha infatti indotto ANAS ad assumere una decisione di tale portata che, seppur penalizzante per il territorio di Lecco e Sondrio, ha sicuramente evitato danni e conseguenze ben più gravi alla galleria e, soprattutto, all'utenza della strada. Il piano alternativo per la viabilità, che in caso di chiusura della strada statale 36 prevede l'utilizzo della strada provinciale 72, è stato immediatamente attivato con l'ausilio delle forze dell'ordine e degli enti locali; la gestione operativa è proseguita con l'intensificazione dell'attività di ANAS che ha garantito il presidio dei punti più critici della viabilità mediante la creazione di otto postazioni fisse lungo la strada provinciale 72. Attualmente, l'attività per il ripristino della viabilità strada statale 36 procede, senza sosta, secondo un cronoprogramma accelerato e concordato tra ANAS e impresa esecutrice dei lavori. descritte, effettuate con turni di 24 ore su 24 e di sette giorni su sette, hanno consentito la riapertura della canna sud della galleria lo scorso 13 giugno, quindi in anticipo rispetto alla precedente previsione del 30 giugno; si renderanno necessarie alcune chiusure notturne della strada statale 36 (tra le ore 22 e le ore 6), per permettere il completamento degli impianti tecnologici e di alcuni lavori di rifinitura, secondo un calendario che verrà definito anche con le amministrazioni locali. I lavori proseguiranno esclusivamente nella canna di monte della galleria con le medesime modalità utilizzate per quella di valle. Le opere, come riferisce ANAS, nonostante le difficoltà intervenute, saranno ultimate nel mese di giugno 2014, grazie all'incremento dei mezzi operativi e delle maestranze, nonché attraverso il potenziamento dei turni lavorativi in modo da accelerare la conclusione Informo, inoltre, che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stanno provvedendo ad effettuare quanto prima, attraverso il provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Lombardia, insieme ad ANAS e agli enti locali interessati, un'accurata verifica della situazione ed un monitoraggio sia da un punto di vista tecnico di sicurezza sia da un punto di vista della sostenibilità nei collegamenti, al fine di migliorare l'attuale situazione critica nei collegamenti stradali della zona. Nel concludere, assicuro che il Governo e il Ministero seguiranno con l'attenzione dovuta, cioè massima, il regolare prosieguo dei lavori.

Signora Presidente, signori del Governo, mi dichiaro soddisfatto della risposta del Sottosegretario, soprattutto per quanto attiene all'attività di vigilanza e monitoraggio per l'immediato ripristino di condizioni di normalità per la viabilità che conduce primariamente in Provincia di Sondrio. detto il Sottosegretario, trattasi di un'arteria strategica che collega Lecco alla Valtellina; forse vale la pena precisare che si tratta fondamentalmente dell'unica che collega un'intera Provincia al resto d'Italia, eccezione fatta per i valichi alpini. A mio avviso, ciò aumenta l'attenzione da parte nostra e del Governo per il futuro, in quanto, nonostante i pronti interventi di ripristino, non possiamo dimenticare che tuttora questa Provincia è collegata solamente con una delle due canne per un importante tratto, proprio quando si sta per inaugurare la strada a quattro corsie in Provincia di Sondrio chiaramente, se l'accesso è ridotto a due corsie, questa importante opera per la nostra Provincia viene fondamentalmente sminuita. Altro motivo di soddisfazione è la vigilanza che il Governo intende assumere riguardo alla cantierizzazione delle opere; non è infatti la prima volta che incidenti di questo tipo capitano su quel tratto. quel tratto. Questi importanti effetti deformanti sono una pericolosa spada di Damocle sull'intera economia della nostra Provincia, per cui si rende necessario capire non solo se vi siano state responsabilità in fase di esecuzione, ma se permangano incognite gravi sul futuro della viabilità di una Provincia vocazione turistica. Occorre capire quindi come attenuare i rischi prevedendo opportuni piani di viabilità alternativa. pur rimarcando che l'azione del Governo non si deve intendere terminata qui, ma che l'importante fase di riscontro, controllo e monitoraggio deve proseguire con maggior insistenza, mi dichiaro soddisfatto.

sia stata sempre piuttosto maldestra per quanto riguarda questa importante arteria. Voglio tuttavia sottolineare il fatto che oggi abbiamo una strada a mezzo servizio. E per il futuro,

isolata dal resto del Paese, perché di fatto è accaduto questo: la Provincia di Sondrio è stata isolata dal resto del Paese, con ricadute devastanti dal punto di vista economico.

non essendo stati chiusi pacchetti turistici importanti per la Provincia, siamo certi di avere un'estate devastante. Allora, signor Sottosegretario, al netto del fatto che abbiamo superato in in questo momento l'emergenza più acuta, quello che chiediamo e su cui vigileremo è che, come promesso dal ministro Lupi e dall'assessore regionale Del Tenno, ci sia un'unione di forze per condividere quello che vuole il territorio, tutti i Comuni rivieraschi, comprese le due Province: la soluzione del peduncolo di Piona, nel dettaglio, e dell'uscita di Dervio. Questo ci darà la garanzia di non essere separati dal resto del Paese. Poi non venite a dire che siamo noi che vogliamo separare il Paese.

dell'interno*. Signora Presidente, l'interrogazione della senatrice Lo Moro richiama l'attenzione del Governo sul ridimensionamento della scorta all'onorevole Angela Napoli, da sempre impegnata nella lotta alla mafia e per l'affermazione della cultura della legalità, chiedendo l'adozione di ogni utile iniziativa volta a ripristinare gli originari dispositivi di sicurezza e di tutela. Innanzitutto, va precisato che le misure di protezione sono adottate a seguito di un'approfondita valutazione della situazione personale di rischio sia in sede locale sia in sede centrale, perché poi possano essere assunte le definitive determinazioni da parte dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. In particolare, per le persone che hanno ricoperto in passato cariche pubbliche, la valutazione sull'effettivo livello di rischio è volta a verificare la qualità o meno dell'esposizione a pericolo. In ogni caso, viene comunque effettuata una periodica e sistematica verifica del grado di personale esposizione al rischio, che costituisce un'ulteriore garanzia dell'effettiva necessità dei servizi di scorta. La materia, peraltro, è stata oggetto di vari correttivi, apportati da ultimo dai decreti del Ministro dell'interno del 23 novembre 2011 e del 3 dicembre 2012, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'uso delle scorte e del contenimento dei costi. Venendo ora allo specifico caso dell'onorevole Napoli, sollevato con l'atto di sindacato ispettivo, preciso che sin dal febbraio 1999 nei confronti dell'ex parlamentare sono stati adottati dispositivi di protezione consistenti in una vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione e la segreteria politica, in quanto la stessa ex parlamentare subiva minacce di morte per la sua attività di denuncia e contrasto alle organizzazioni criminali calabresi. A partire dal 1992, in funzione degli incarichi istituzionali svolti e di alcuni episodi intimidatori, sono state disposte più incisive misure di protezione, e da ultimo è stato disposto un servizio di scorta di cosiddetto terzo livello. Lo scorso 6 maggio, in sede di revisione periodica dei dispositivi di tutela e in considerazione della cessazione delle funzioni parlamentari, è stata disposta la rimodulazione della misura nel quarto livello. Sulla base però delle preoccupazioni emerse in merito alla sicurezza personale dell'interessata, la situazione è stata riesaminata dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza, che ha disposto il ripristino, come peraltro richiesto dalla senatrice Lo Moro con la sua interrogazione,

Noi siamo intervenuti tempestivamente, perché ci sembrava doveroso, nel momento in cui c'è stato un cambio di Governo e la cosa poteva non essere evidenziata in maniera adeguata, segnalare un caso che per chi vive in Calabria era di autentico pericolo. Non basta la cessazione di un'attività per porre fine a un pericolo. Quando si fa sul serio il parlamentare, quando si fa politica, anche senza essere parlamentare, quando si è militanti dell'antimafia, come è stata a lungo e continua ad essere Angela Napoli, bisogna essere più cauti. Naturalmente non mi sto riferendo a lei e al suo Governo, vice ministro Bubbico, perché tra l'altro non siete voi i destinatari di alcuna recriminazione. Però questo caso ci fa riflettere. Ci fa riflettere sui momenti delicati di passaggio. Ci fa riflettere sulle strutture. Ci fa riflettere sulla visione che hanno le strutture

fare questa osservazione. Ringrazio per la tempestività, ma quel che è successo deve servire a guidarci per il futuro, perché le situazioni vanno riviste ciclicamente. Lo dico subito e lo dico chiaro: non sono per le scorte utilizzate come *status symbol*, anzi sono proprio contraria a questo modo di manifestare e di rappresentare il proprio ruolo. Ma quando le scorte sono giustificate da pericoli reali vanno assegnate e mantenute. Soprattutto, non si può lasciare sola da un momento all'altro una persona,

Signor Presidente, onorevoli senatori, la disciplina dell'assunzione di personale nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato è regolata dal codice dell'ordinamento militare, che prevede l'osservanza di procedure e modalità operative cui l'amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta a conformarsi. La normativa in vigore stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, come per le altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nella carriera iniziale della Polizia di Stato vengano determinati sulla base di una «programmazione quinquennale scorrevole». Questi programmi, annualmente predisposti da ciascuna delle amministrazioni interessate, sono comunicati entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero della difesa. I posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale. Solo il 55 per cento dei concorrenti giudicati idonei dopo almeno un anno di servizio svolto presso le Forze armate ed utilmente collocati nelle graduatorie viene immesso direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia. Il restante 45 può essere invece immesso in ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma permanente quadriennale. L'amministrazione della Pubblica sicurezza, pertanto, è obbligata al rispetto del procedimento concorsuale previsto dalla normativa di settore che consente l'immissione nel ruolo iniziale della Polizia di Stato solo dopo lo svolgimento dei quattro anni di ferma. D'altra parte, bisogna anche tener conto che la stessa disciplina normativa richiede che venga effettuata con periodicità l'attività concorsuale, bandendo nuove procedure selettive anche per far fronte alle esigenze di personale delle strutture militari. Ricordo anche che la legge di stabilità per il 2013, relativamente alle assunzioni nelle Forze di polizia e disciplina del *turnover*, ha previsto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dal 2014, fondi che permetteranno alle amministrazioni interessate di avere un margine più agevole di manovra nelle facoltà di assunzione, anche relativamente ai volontari in ferma prefissata.

purtroppo a nascondersi dietro fantasiose esigenze di cassa, quasi consapevolmente ignaro che solo la soluzione che proponiamo da un anno è orientata al reale risparmio. È come se la macchina amministrativa, arrivata ad un certo punto, si inceppasse e non fosse più capace di operare scelte diverse. Di recente anche i *media* hanno dato risalto alla questione delle seconde aliquote, dando voce e riportando all'attenzione dell'opinione pubblica un dramma che non riguarda genericamente gli sprechi della pubblica amministrazione, ma nello specifico la vita, i sogni e le aspettative di 1.700 ragazzi. Da un anno cerco di elevare l'attenzione del suo Ministero nei confronti di questa questione. Ci sono stati momenti di incontro, atti di sindacato ispettivo, proposte emendative, che si sono però limitati a impegni di natura politica e si sono tradotti soltanto in un allentamento delle maglie del *turnover* nel comparto della sicurezza e della difesa. Questa premessa è certamente necessaria per il reintegro dei vincitori di concorso posti in seconda aliquota, ma appare opportuno segnalare che su questo argomento non bisogna attendere di convincere questo o quello per ottenere qualche risultato: bisognerebbe soltanto essere razionali tutti insieme e capire che, dietro certe leggi, si nascondono spesso esigenze assurde. Con questo non voglio addebitare a lei o all'attuale Ministro, essendo in carica da pochi mesi, quel mal sistema che è andato sedimentandosi in questi sette anni, che non considera che molti ragazzi stanno affrontando un percorso a ostacoli, spesso rinunciando al progetto di mettersi al servizio del loro Paese. Non le nego, signor Vice Ministro, che mi ha particolarmente confuso l'indizione di un nuovo concorso lo scorso mese di marzo per il reclutamento di 964 allievi agenti. Cosa c'entra un nuovo concorso, mentre altri 1.700 ragazzi attendono da anni? A parte il non trascurabile spreco di risorse, questo intervento vanifica la prospettiva di ammissione nella carriera iniziale dei giovani vincitori di concorso, oltre a contraddire quanto previsto dalla normativa e dai requisiti dei concorsi a cui i giovani hanno preso parte.

a sperare di entrare a 30 anni, con ovvie conseguenze in termini di operatività e di efficienza delle nostre forze dell'ordine. Signor Vice Ministro, il punto su cui concentrarsi è uno solo: per far fronte al fabbisogno di personale tutte le amministrazioni dovrebbero utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già svolti e assolutamente non indire nuovi concorsi. Dobbiamo mettere la parola fine al solito sistema Italia, dove, invece di trovare le soluzioni più semplici e fattibili, si complica tutto perché non si ha una visione strategica. Questa è la vera *spending* *review*, attraverso la quale da un lato si riducono le spese e, dall'altro, si colma un *vulnus* normativo pesante. Deve essere inderogabile consentire l'entrata dei vincitori dei primi concorsi della Polizia di Stato, mettendo in atto tutte le procedure amministrative necessarie prima che si concluda il servizio nelle Forze armate, al fine di evitare che questi giovani rimangano anche senza lavoro, in attesa di transitare nella Polizia. Inoltre, è necessario - e sono certo che il Ministero se ne prenderà l'incarico - avviare la modifica della norma vigente al fine di depennare la disciplina, mettendo in *stand

dove si assiste ad una crescita dei reati che genera un senso di insicurezza tra i cittadini, il mantenimento di questo *status quo* rischia di essere particolarmente deleterio. Concludo, signora Presidente. Abbiamo l'esigenza di ridare dignità a

che è legata alla signora Annunziata Vagnoni, dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che appartiene alla prima area funzionale, fascia retributiva F2, con la qualifica di collaboratore scolastico a tempo indeterminato presso l'Istituto comprensivo «G. Leopardi» di Grottammare, in Provincia di Ascoli. La signora presta servizio a titolo di comando presso l'Archivio di Stato di Fermo e, pur se inquadrata in quest'area prima, possiede requisiti culturali e capacità operativa per assicurare il regolare andamento dei servizi al pubblico e il supporto al direttore nella sua attività tecnico-scientifica. Lo scorso anno, purtroppo, in occasione della decisione di revoca del comando avanzata dalla sua amministrazione di origine (il MIUR), questo Ministero era intervenuto presso il competente ufficio scolastico regionale per ottenere la sospensione della revoca del comando e scongiurare il conseguente richiamo della collaboratrice nell'amministrazione di appartenenza. Questo Ministero ha dovuto, invece, procedere comunque alla revoca del comando della dipendente in argomento, analogamente con quanto disposto in altri tredici casi simili, l'8 marzo 2013, con con provvedimento della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, perché nel frattempo era stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il 22 gennaio 2013, che approvava la nuova dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali. A seguito di tale ridimensionamento, la pianta organica di questo Ministero, come correttamente da lei riferito nella sua interrogazione, senatore Verducci, prevede ora soltanto 700 posti in prima area.

Ma la permanenza di dipendenti in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni presuppone la disponibilità di posti in organico, che, nel caso di specie, non era più sussistente in prima area, a seguito dell'emanazione del citato Il direttore dell'Archivio di Stato di Fermo non ha mancato di segnalare le ricadute negative di questa revoca sul regolare andamento dell'istituto e sull'immagine pubblica del Ministero. Analoghe preoccupazioni sono state espresse dal direttore generale delle Marche, dall'amministrazione provinciale di Fermo, dall'Università di Macerata e dalla stessa Direzione generale degli archivi. Purtroppo, non abbiamo potuto che ribadire, allo stato attuale della normativa, l'operato dell'amministrazione, anche in considerazione dei numerosi richiami che sono stati formulati dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero in merito all'esigenza di verificare puntualmente la capienza di posti in organico all'interno delle aree prima di mantenere in servizio il personale comandato.

non possono indurmi ad esprimere soddisfazione quanto - piuttosto - ad aumentare il rammarico per una norma che rischia di compromettere la funzionalità dei nostri archivi. Signora Sottosegretario, mi rifaccio alla conclusione del suo intervento per invitare davvero e in maniera pressante il Governo ad accendere i riflettori su questa realtà (non solo su quella specifica richiamata dall'interrogazione) e fare in modo che la funzionalità dei nostri archivi non venga compromessa. È chiaro che questa interrogazione nasce da un caso specifico e urgente, che lei richiamava, ma nel depositarla ho voluto rimarcare anche i tratti della sua emblematicità: il caso specifico di Fermo è in realtà il caso dell'intero sistema diffuso degli archivi e - potrei aggiungere - delle biblioteche nel nostro Paese, le cui funzionalità e potenzialità sono letteralmente inibite da tagli che in questi anni sono stati continui e pesantissimi e da una cronica carenza di personale, acuita molto gravemente dai cosiddetti provvedimenti di *spending review*.

a tutti i livelli. Questo è dovuto alle caratteristiche del nostro sistema policentrico e alla cultura delle nostre autonomie. Pertanto, quando noi mettiamo a rischio la funzionalità di un archivio e il suo rapporto con la comunità locale degli studi, a partire dagli studenti, non solo mettiamo a rischio la

Per questo non possiamo tollerare la pessima condizione dell'edilizia archivistica: molto spesso ci sono archivi interi ridotti a scantinati o situati in luoghi non adatti. Non possiamo neanche tollerare che il personale degli archivi debba combattere con un sottodimensionamento ormai cronico. Eppure sono figure professionali di altissimo livello, che necessitano di anni per formarsi e la cui competenza non si esaurisce nel solo percorso scolastico-universitario. Sarebbe urgente, ad esempio, indire un concorso per giovani archivisti: non è indetto da decenni. Parimenti non sono più tollerabili forme contrattuali troppo precarie. Dobbiamo inoltre rilanciare il ruolo dell'Italia nei comitati internazionali, nei quali è unanimemente riconosciuta la qualità e la competenza dei nostri archivisti. Signora rappresentante del Governo, dovremmo intervenire sul piano normativo e inserire nel codice dei beni culturali un capitolo specifico dedicato ad archivi e biblioteche e fare in modo che esse appartengano al al patrimonio culturale del nostro Paese. Ci interroghiamo molto spesso in questi tempi di crisi su quale sia il ruolo del nostro Paese nel mondo: io penso che esso abbia a che fare con la forza della nostra identità, con la sua riconoscibilità che contraddistingue la forza culturale, prima che commerciale, del nostro *made in Italy*. Di tutto questo, al fondo, tratta questa interrogazione così urgente.

impone alcune riflessioni in ordine alla qualità e alle modalità di trasmissione del servizio pubblico televisivo. Il dottor Angelo Di Natale da anni denuncia una serie di episodi e comportamenti che gettano un'ombra preoccupante sulla gestione dell'informazione pubblica, quanto meno all'interno della redazione RAI di Catania. A fronte di tali reiterate e circostanziate denunce, la risposta dell'azienda è stata sbrigativa nell'accertamento, ma molto reattiva e sanzionatoria nei confronti del denunciante che, dopo aver scontato varie sospensioni dal servizio, si vede oggi applicata una sanzione ampiamente spropositata. Licenziare in tronco un dipendente che denuncia gravi comportamenti nella gestione di un delicatissimo servizio qual è la pubblica informazione appare un atto obiettivamente minaccioso e ammonitorio nei confronti degli altri dipendenti. Fatte salve le opportune verifiche da parte degli organi competenti, i gravi fatti denunciati dal dottor Di Natale meritano approfondimenti e indagini incisive ed esaurienti a tutela dell'immagine della RAI. Il Movimento 5 Stelle, nell'affermare la solidarietà e la vicinanza nei confronti dei giornalisti che credono nel diritto e dovere di informare con responsabilità e libertà, continuerà a combattere ogni forma distorsiva del servizio di informazione generale. Siamo convinti che l'informazione debba essere critica e libera da condizionamenti di qualsiasi natura e per tale motivo difenderemo i principi di verità, responsabilità, etica e deontologia professionale giornalistica oltre che i doveri del servizio pubblico dell'informazione,